all'apertura, appunto, dei nostri lavori. Noi non possiamo far finta che non sia accaduto nulla, signor Presidente, e neanche vogliamo enfatizzare quello che è accaduto; vogliamo però, realisticamente, ricordare a noi stessi meno di due ore fa, il Governo non ha ottenuto la maggioranza in quest'Aula in un momento molto difficile, molto delicato, perché il fatto che quanto dichiarato dal ministro D'Alema non sia stato accolto dalla maggioranza dei senatori, documentando così l'assenza di una maggioranza reale di sostegno al Governo,

non c'era la maggioranza - parlo della relazione del ministro della difesa Parisi - e, di conseguenza, c'è stata questa necessità, ritengo voluta anche da parte del Presidente della Repubblica, di verificare se al Senato vi fosse o non vi fosse una maggioranza reale a sostegno del Governo. Ebbene, oggi è stato dimostrato, confermato che sulla politica estera

che, mentre ci sono incontri e si prevede già per questa sera, alle ore 19, l'incontro del Presidente del Consiglio con il Presidente della Repubblica, noi non possiamo continuare a discutere e a parlare come se nulla

assolutamente consci dell'importanza del disegno di legge *in* *itinere*, riteniamo che questo sia un momento talmente difficile da dover essere oggetto di chiarificazione e pertanto dobbiamo avere rispetto per gli organi superiori.

in questa sede, di maramaldeggiare e quindi non farò considerazioni di questa natura, tuttavia, un dato non può sfuggire: oggi, su tutti i giornali,

Prendendo atto di quanto affermato dal Ministro degli affari esteri, ne deriva immancabilmente che in questo momento non abbiamo più un Governo, anche se da un punto di vista meramente formale e costituzionale è ancora in piedi. D'altro canto, mi pare che, *ictu oculi,*

i Gruppi hanno già espresso la loro opinione e pertanto non possiamo che ripetere le argomentazioni che sono già state svolte. Il Presidente della nostra Assemblea ha giustamente concluso che i lavori sarebbero ripresi e che avrebbe seguito il calendario. Io non posso che ricordare alla Presidenza e soprattutto ai colleghi dell'opposizione che quel che è accaduto è accaduto; questa sera ci sarà la Conferenza dei Capigruppo; il Consiglio dei ministri prenderà le sue decisioni; il Presidente della Repubblica, investito

atteso che il Presidente del Senato aveva già risposto a queste argomentazioni dicendo che avremmo ripreso, riteniamo che si debba proseguire nei nostri lavori, anche per senso di responsabilità, Presidente, perché quello che può accadere potrebbe poi fermare non per un'ora o un giorno, ma magari per più tempo i lavori, e ci troveremmo con un decreto non convertito, che pure contiene materie di un certo interesse, e a non discutere una proposta di legge sulla quale vi è una larga convergenza che risolverebbe dei problemi. Per senso di responsabilità e anche per continuità dell'azione delle istituzioni, noi riteniamo ci siano le condizioni per andare avanti.

mi associo a quanto appena detto dal senatore Boccia, sottolineando anche il fatto, già rilevato una volta, che quanto successo è sicuramente un fatto politico rilevante, ma non è una crisi di Governo che deve seguire la

e segnatamente con gli articoli che disciplinano il sistema e la regolarità delle votazioni. Poiché questa mattina si è parlato molto di guerra preventiva, io ho necessità di far capire al collega Boccia che vanno comprese le ragioni dell'opposizione che in quest'Aula è diventata maggioranza.

la cosa più importante è la politica estera. Qui vi è stata una sfida all'opposizione. La mattina ci si è travestiti con un ragionamento forlaniano; poi si è indossata la divisa togliattiana; infine, si è finiti come Comunardo Niccolai con un autogol. E adesso ci venite a chiedere il senso di responsabilità. Perché un richiamo al Regolamento? Perché così ci costringete a dover chiedere la verifica del numero legale sin dal primo articolo e su questo ci bloccheremo. Allora, prudenza vuole che si accolga il suggerimento del collega Tofani, non credo che riuscirete a mobilitare senatori a vita, deputati a vita e chissà quanti altri per mantenere il numero legale in quest'Aula. La figura meritata che avete fatto oggi, grazie all'arroganza del Ministro degli affari esteri, non pensate di farla passare inosservata e poter andare avanti come se nulla fosse

Presidente, non aggiungo molto a quanto affermato dal senatore Boccia, che condivido. Desidero solo segnalare il fatto che

A norma di Regolamento avrei dovuto far parlare un senatore a favore e uno contro; data la particolare e specifica situazione che stiamo vivendo, ho ritenuto opportuno sentire in Aula i rappresentanti sia dell'opposizione che della maggioranza.

mi sembra ragionevole e che potrebbe, non dico vanificare quella richiesta di votazione, ma quantomeno differirla. È vero che abbiamo all'ordine del giorno un decreto‑legge che scade fra quattro giorni, però, è pur vero che abbiamo anche un altro provvedimento

signor Presidente, chiedo formalmente un'inversione dell'ordine del giorno per poter trattare prima la richiesta di costituzione in giudizio per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal GIP di Milano nei confronti del Senato con riferimento ad una dichiarazione di insindacabilità

anche noi siamo d'accordo con la proposta del collega Manzione ad una condizione, che riteniamo molto importante, e cioè che si proceda solo con quel provvedimento al quale ha fatto riferimento il collega Manzione.

- ma forse molti colleghi lo sanno - che il Presidente del Consiglio si recherà, alle ore 19, presso il Quirinale. Comunico, altresì, che è stata convocata per le ore 18, qui in Senato, la Conferenza dei Capigruppo.

Con ricorso del 22 luglio 2006, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale, il tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta 18 gennaio 2006, ha dichiarato che i fatti oggetto del procedimento penale n. 5813/05 RGNR - n. 4741/05 RG GIP, pendente nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili ai sensi dell'articolo Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 10 gennaio 2007, n. 17, depositata in cancelleria il successivo 26 gennaio e notificata al Senato il 12 febbraio 2007. Nella seduta odierna la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, all'unanimità, nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto. Se l'Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

ancora una volta quest'Aula è chiamata a decidere in merito ad un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, sollevato dal potere cosiddetto giudiziario nei confronti del Parlamento e, nella specie, del Senato. Il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, nel caso di specie, è stato sollevato dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale iscritto presso quella sede giudiziaria e pendente davanti al GIP di quel tribunale. *(Brusìo).* Se i colleghi mi consentono di parlare, li ringrazio.

In merito a questo procedimento vi è stata, da parte del Senato della Repubblica, una deliberazione, datata 18 gennaio 2006, in forza della quale è stata riconosciuta l'insindacabilità dei comportamenti del collega Iannuzzi, proprio relativamente al procedimento penale che ho indicato poc'anzi. Il tutto traeva origine da presunte offese arrecate alla reputazione di Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte, alla pubblicazione sul quotidiano «il Giornale» del 7 novembre 2004 di un articolo intitolato «Mafia, 13 anni di scontri fra PM e Carabinieri». il Senato della Repubblica ha ritenuto sussistere l'esimente di cui all'articolo 68 della Costituzione, ma, com'è previsto, il GIP presso il tribunale di Milano, ritenendo che il Senato, in qualche modo, fosse andato oltre i limiti di applicabilità del suddetto articolo, ha sollevato il conflitto di attribuzione. La Corte costituzionale, signor Presidente, ha ritenuto ammissibile - come ella ha ricordato poco fa - il ricorso e, quindi, adesso è necessario decidere se costituirsi oppure no in giudizio per resistere nel conflitto di attribuzione alle richieste avanzate dal GIP di Milano. Come mi è già capitato di fare in quest'Aula (molto più tranquilla in altre occasioni, anche se molto più affollata), pur avendo votato contro la richiesta di applicazione dell'articolo 68 in favore del collega Lino Iannuzzi nella seduta del 18 gennaio 2006 (quindi, avendo espresso, nel merito, un voto contrario), ritengo che il Senato sia obbligato a coltivare la costituzione in giudizio. Non a caso ribadisco che, molto spesso, in questi casi - e chiedo scusa ai colleghi che sono costretti ad ascoltare sempre la stessa argomentazione, però è giusto che resti, comunque, agli atti - posso non condividere una proposta di legge, ma, nel momento in cui legittimamente il Parlamento la approva, essa, una volta divenuta legge, è vincolante per tutti, anche per chi, in quel momento, credeva una cosa diversa.

la volontà di un organo di rango costituzionale. In questa logica, pur essendomi espresso nel merito contro, ritengo che il Senato sia obbligato a costituirsi in giudizio per coltivare le difese che riterrà opportune proprio all'interno del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal GIP di Milano. In questa logica, concludo affinché il Senato voglia conseguentemente

finestra"). Metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relative alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano. **Sono approvate.** La Presidenza tribunale di Milano. **Sono approvate.** La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.